L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.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 Comunico che in data 8 ottobre è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri della salute, della cultura, dello sviluppo economico, dell'interno e della giustizia:* «Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali,

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario della settimana corrente e il nuovo calendario dei lavori L'ordine del giorno della seduta di oggi prevede la discussione del decreto-legge sulla crisi d'impresa. Il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia su un emendamento interamente sostitutivo del provvedimento. Si è stabilito che le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia avranno luogo nella seduta di domani, a partire dalle ore 9,30. Seguirà la chiama. Successivamente sarà discusso il decreto-legge sulle modalità operative relative alle consultazioni elettorali 2021, già approvato dalla Camera dei deputati. Gli emendamenti a tale decreto dovranno essere presentati oggi, entro le ore 18. oggi, entro le ore 18. Sempre nella seduta di domani saranno esaminati il disegno di legge recante l'intesa con l'associazione Chiesa d'Inghilterra e i disegni di legge recanti ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri. Martedì 19 ottobre, alle ore 16,30, il Ministro dell'interno renderà - come richiesto - un'informativa sui gravi fatti accaduti a Roma il 9 ottobre in occasione della manifestazione svoltasi presso piazza del Popolo. Seguirà l'eventuale esame di ratifiche non discusse nella seduta di domani. Restano confermate, per mercoledì 20 ottobre, alle ore 9, le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre 2021. Nel pomeriggio di mercoledì 20, alle ore 14,30, saranno discusse mozioni su iniziative volte a dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e mozioni su iniziative volte a contrastare ogni forma di violenza e di totalitarismo, i cui testi dovranno pervenire entro le ore 12 di martedì 19 ottobre. La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi nella stessa giornata di martedì 19, alle ore 15, per definire l'ulteriore programmazione dei lavori.

Presidente, Governo, sottosegretario Sisto, colleghi, questo decreto-legge, che è stato ampiamente modificato in Commissione, si compone di due parti: la prima riguarda la crisi d'impresa, mentre la seconda reca misure urgenti in materia di giustizia.

Tale quadro va rinvenuto nelle dichiarazioni che fece il presidente Draghi quando venne in Parlamento a chiedere la fiducia

si inquadrano in un disegno più ampio, che riguarda la riforma del processo civile, che questa Assemblea ha recentemente approvato,

e tutta la partita che ha ad oggetto il codice dell'insolvenza e della crisi d'impresa. Senza questi riferimenti è difficile capire capire perché oggi si parla con urgenza di crisi d'impresa e di giustizia. In modo particolare dobbiamo tenere conto del

le risoluzioni extragiudiziarie), i meccanismi di allerta, la specializzazione degli uffici giudiziari e la creazione di piattaforme *online*. Su queste riforme ha operato una commissione ministeriale, la commissione Pagni;

- ha come obiettivo principale la garanzia, per le imprese e gli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie, finanziarie, di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, gli imprenditori onesti ma insolventi o sopra indebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante anche l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo e di conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione anche attraverso la riduzione della loro durata. Tutto ciò è importante perché in più occasioni ci siamo chiesti che fine avrebbero fatto le aziende colpite duramente dalla crisi economica per il Covid-19 e che magari lo erano già prima

negoziata della crisi. In pratica, su impulso dell'imprenditore - è l'imprenditore in primo luogo che si muove - si cerca un risanamento naturalmente si dà la possibilità di avere un supporto attraverso degli esperti, che lo affiancano ma non lo sostituiscono, attraverso la piattaforma che è già in opera fatta con le camere di commercio, attraverso misure protettive che riguardano tutti i crediti che coinvolgono i diritti del lavoratore

Questo impianto consente all'imprenditore con una procedura negoziale volontaria di chiudere un contratto con uno o più creditori, di fare una convenzione di moratoria, di chiudere un accordo con tutti, di ristrutturare il debito oppure di fare un piano di risanamento, un concordato semplificato per esempio, l'amministrazione straordinaria, se parliamo di grandi imprese, con dei benefici da una parte di carattere fiscale e, dall'altra, delle misure di protezione. Per esempio, penso alla bancarotta fraudolenta e semplice. alla traduzione operativa. È una materia che può sembrare molto tecnica e complessa, ma in realtà è una chiave di volta a fronte di una situazione come quella che viviamo,

l'aumento dell'organico di 20 magistrati per coprire il buco che si è creato con la procura europea e soprattutto un concorso per coprire i posti vacanti per 500 magistrati, misura che si collega evidentemente a tutti i ragionamenti che ci sono stati soprattutto in sede di approvazione della delega civile,

*relatore*. Signor Presidente, colleghi, le Commissioni riunite 2a e 10a hanno svolto un proficuo lavoro di rafforzamento del provvedimento in esame attraverso l'approvazione di emendamenti migliorativi, frutto di una fattiva collaborazione tra Governo e forze di maggioranza. Un pacchetto consistente di modifiche ha riguardato proprio la composizione negoziata per la soluzione delle crisi di impresa. Le Commissioni hanno provveduto a un'integrale sostituzione dell'articolo 3. Rispetto al testo originale il nuovo articolo prevede numerose innovazioni a cominciare dal potenziamento della piattaforma telematica. Nella nuova formulazione essa è gestita dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico. Essa inoltre rende disponibile anche un protocollo di conduzione della composizione negoziata. Si prevede inoltre esplicitamente di adeguare la lista di controllo anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese. Anche le procedure vengono migliorate - ad esempio - rendendo più flessibile il ricorso a commercialisti ed esperti contabili; prevedendo un coinvolgimento maggiore degli ordini professionali di appartenenza dei professionisti e dando maggiore flessibilità temporale al segretario generale della camera di commercio nella comunicazione alla Commissione. Viene infine data maggiore importanza all'esperienza formativa dei professionisti nelle materie rilevanti, come risulta dal *curriculum*. Con le modifiche all'articolo 4 vengono rafforzati i requisiti di indipendenza delle persone che svolgono incarichi nelle procedure previste dal decreto-legge in esame; in esame; gli esperti non possono intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata e devono risultare terzi rispetto a tutte le parti. All'articolo 5 sono portati miglioramenti all'accesso alla composizione negoziata; innanzitutto all'imprenditore viene richiesto di inserire nella banca dati telematica anche una dichiarazione con la quale attesta di non aver depositato determinati ricorsi. Inoltre, il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi non può essere sostituito, se non disponibile, dal documento unico di regolarità contributiva. Anche all'articolo 5 si rafforzano i requisiti dell'incarico dell'esperto; non possono superare i centottanta giorni, ma con una formulazione più forte del testo originale si può proseguire per altri centottanta giorni con il consenso di tutte le parti. All'articolo 6 vi sono le modifiche specifiche ai crediti anteriori, il cui mancato pagamento impedisce il rifiuto dell'adempimento della risoluzione dei contratti pendenti da parte dei creditori interessati dalle misure protettive che sono anteriori alla pubblicazione dell'istanza. All'articolo 7 si specifica che il giorno della presentazione del ricorso è lo stesso della pubblicazione della richiesta dell'accettazione dell'esperto. All'articolo 8 è prevista una nuova possibilità per l'imprenditore, il quale può dichiarare che non si applicano su di lui gli obblighi di riduzione del capitale per perdite di riduzione dei capitali sociali, di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile, anche con dichiarazione effettuata tramite la piattaforma telematica e pubblicata nel registro delle imprese, momento in cui gli effetti della dichiarazione o dell'istanza entrano in vigore. All'articolo 9 si specifica la condotta dell'imprenditore. A lui è chiesto di gestire l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività, non solo quando sussiste probabilità di insolvenza. Quando sussiste tale probabilità, ma con concrete prospettive di risanamento, l'imprenditore gestisce l'attività nel prevalente interesse dei creditori, restando ferme le sue responsabilità. Si stabilisce, all'articolo 10, che l'autorizzazione all'imprenditore per la cessione dell'azienda da parte del tribunale avviene dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti. All'articolo 11 vengono apportati tre miglioramenti. Innanzitutto, viene riformulata la norma sulla non necessarietà dell'attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano di risanamento. L'imprenditore, inoltre, può proporre la domanda di concordato semplificato solo all'esito delle trattative e, infine, si introduce una norma specifica per le imprese agricole, le quali possono, in alternativa alle soluzioni proposte, accedere alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni disciplinati dagli articoli 7 e 14-*ter* della legge 27 gennaio 2012, n. 3. Passando all'articolo 15, un emendamento approvato elimina possibili dubbi interpretativi grazie alla disposizione vigente, in ragione della natura solidale della responsabilità dei sindaci rispetto a quella dell'organo amministrativo. L'articolo 16 viene rafforzato prevedendo nuove modalità di determinazione del compenso dell'esperto, al fine di incentivare quanto più possibile gli esiti preferibili. All'articolo 17 si amplia la documentazione che l'imprenditore sotto soglia deve produrre al fine di esentare l'esperto dall'acquisizione della documentazione contabile dell'impresa e dalla redazione della relazione sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'imprenditore e dall'elenco aggiornato dei creditori dei relativi diritti, trattandosi di attività particolarmente onerose, non compatibili con la speditezza della composizione. Per quanto riguarda l'articolo 18, vengono arricchite le condizioni per l'accesso al concordato semplificato, al fine di collegare tale opzione al regolare e corretto svolgimento delle trattative e di prevenire condotte abusive. All'articolo 20, tra i presupposti degli accordi ad efficacia estesa, è precisato che la soddisfazione dei creditori deve essere garantita in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria, cioè rispetto all'alternativa del fallimento, secondo quanto previsto dalla analoga disposizione presente nel codice della crisi d'impresa, all'articolo 61, Inoltre, nel sancire l'indifferenza dell'accordo rispetto alle ipoteche iscritte nei novanta giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese, si incentiva il ricorso a tale strumento di composizione negoziata della crisi. Le ultime modifiche approvate riguardano l'articolo 23. L'istanza di composizione negoziata non può essere presentata in presenza di procedimento con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 182-*bis*, sesto comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o con ricorso per l'accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 14-*ter* della legge 27 gennaio 2012, n. 3. Infine, è previsto che le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, si applicano a tutte le procedure concorsuali e ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti. interventi aggiuntivi sono stati già descritti dalla relatrice Modena. Io aggiungo solamente, in conclusione, che quello in esame è un provvedimento significativo, che sicuramente aiuterà le imprese in questa fase di rilancio dell'economia e che sicuramente porta con sé tante contraddizioni in uscita dalla pandemia. Certamente, la nuova procedura dovrà essere rivista e valutata, anche a seguito dei dati che ci perverranno nella sua applicazione, per capire, nel momento in cui non non sarà più possibile prorogare l'entrata in vigore del codice di crisi, che tipo di rapporto ci sarà tra queste due procedure. Chiaramente, questa è una nuova procedura inserita in attesa che entri in vigore il codice di crisi. Quando entrerà in vigore il codice di crisi, dovremo fare le valutazioni su come la nuova procedura potrà essere eventualmente proseguita o implementata in modo differente.

le disposizioni del presente testo nascono dalla necessità d'intervenire nell'attuale contesto socio-economico per contrastare gli effetti che la crisi ha prodotto nelle imprese e il sovraindebitamento, intervenendo in tema di insolvenza e delle procedure concorsuali ad essa relative, al fine di individuare misure idonee ad incentivare l'emersione dalla crisi in un periodo temporale così delicato, che mina seriamente le dinamiche produttive con risvolti molto seri sotto il profilo occupazionale e che aggrediscono il ciclo produttivo di gran parte dell'economia nazionale. Vari provvedimenti a carattere straordinario ed emergenziale si sono susseguiti nel corso di questo periodo, periodo, con diversi obiettivi di tutela della salute pubblica, dell'occupazione, del tessuto economico e sociale generale. Tuttavia, altri e diversi diversi strumenti devono apprestarsi nel momento di transizione in una fase di ripresa, come quella attuale, per sollecitare lo sviluppo in tutti i settori. È a questo punto che possono prospettarsi diversi scenari, da una situazione di crisi di liquidità temporanea e irreversibile sino alle più gravi situazioni di perdita della continuità aziendale stessa, nonché di crisi o insolvenza dell'impresa. La prospettiva delineata ha fatto considerare l'entrata in vigore il 15 agosto 2020 del decreto legislativo n. 14 del 2019, che già prevedeva la riforma del diritto fallimentare attraverso l'introduzione del codice della crisi, in cui vengono individuati meccanismi di risoluzione alternativi delle crisi, nonché strumenti di allerta che prodromicamente consentono di intervenire per mitigare gli effetti dell'indebitamento, permettendo continuità dell'attività aziendale tramite soluzioni anche stragiudiziali. In caso contrario sono favorite procedure semplificate di cessazione dell'azienda o di ramo della stessa. Tuttavia, l'entrata in vigore del codice avrebbe determinato l'abrogazione dell'attuale legge fallimentare, con la conseguenza che un numero elevato di casi di crisi d'impresa, gran parte dei quali diretta conseguenza del Covid, sarebbero stati regolati da un corpo normativo del tutto nuovo. Per evitare, quindi, che le incertezze applicative della disciplina o il funzionamento di istituti discussi, quali le misure di allerta, potessero aggravare ulteriormente la situazione di difficoltà delle imprese, l'articolo 5 del decreto-legge liquidità aveva opportunamente rinviato il termine di entrata in vigore del complesso normativo intero al primo settembre 2021. Il decreto-legge in esame reca misure urgenti in materia di crisi d'impresa e risanamento aziendale e prevede ulteriori misure urgenti anche in materia di giustizia. In particolare, rinvia l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza al 16 maggio 2022, ad eccezione di disposizioni di cui a un titolo specifico del codice (il secondo), concernenti le procedure di allerta e la composizione assistita della crisi innanzi a un organismo di composizione della crisi di impresa (Ocri), per le quali l'entrata in vigore è fissata al 31 introduce e disciplina, in particolare, la procedura di composizione negoziata della crisi: un nuovo istituto volontario cui si accede tramite una istituenda piattaforma telematica nazionale, che offre all'imprenditore l'affiancamento di un esperto terzo e indipendente per agevolare, in maniera anche riservata, le trattative con i creditori. Il decreto-legge disciplina nel dettaglio possibili soluzioni adottabili in esito alla procedura e prevede, tra l'altro, nel caso di mancata individuazione di una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi, la possibilità per l'imprenditore di presentare una proposta di concordato per cessione di beni, unitamente al piano di liquidazione, il cosiddetto concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Il testo apporta una serie di modifiche anche alla legge fallimentare, con l'anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale previsti dal codice della crisi. Dispone, tra l'altro - e questo è importante - un aumento di venti unità nel ruolo organico del personale della magistratura ordinaria, troppo spesso in sofferenza, al fine di garantire che l'attuazione che l'attuazione della normativa europea relativa alla procura europea istituita, e in virtù della quale sono stati attribuiti a venti magistrati funzioni di procuratore europeo delegato, non privi di risorse la magistratura e le procure della Repubblica. testo reca anche misure volte ad accelerare, attraverso il ricorso alla digitalizzazione, le procedure di pagamento degli indennizzi per la equa riparazione, in caso di violazione del termine della ragionevole durata del processo - un altro tema centrale del nostro sistema giustizia - e delle altre somme dovute sulla base dei titoli giudiziari. Introduce una disciplina derogatoria, valida soltanto per l'anno 2021, in materia di assegnazione di risorse del Fondo unico di giustizia (FUG), prevedendo la riassegnazione immediata delle quote versate all'entrata di bilancio dello Stato nel 2020 e agli atti di previsione dei Ministeri della giustizia e dell'interno. In corso di esame nelle Commissioni riunite, che ringrazio per il pregevole contributo, sono state introdotte significative proposte emendative: in particolare, appare di pregio la riscrittura dell'articolo 3, proposta con un apposito emendamento, con cui si specifica che la piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico, intervenendo sulle modalità di iscrizione all'elenco degli esperti. Vi è poi l'inserimento, proposto con un apposito emendamento, di specifiche disposizioni in materia di procedure di amministrazione straordinaria per le grandi imprese insolventi, l'introduzione di specifiche disposizioni in materia di concorso per il reclutamento di magistrati ordinari, tema quest'ultimo molto significativo. Nel settore della giustizia,

lo stesso Consiglio europeo, nelle annuali raccomandazioni che sovente anticipano ogni atto, in particolare della 2a Commissione, ha sollecitato l'Italia a ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio, nonché ad aumentare l'efficacia della prevenzione e repressione della corruzione, riducendo la durata dei processi penali e attuando il nuovo quadro anticorruzione. Lo stesso PNRR individua nella lentezza della realizzazione di alcune riforme strutturali un limite potenziale di crescita del nostro Paese. Per raggiungere questi obiettivi, quindi, gli ambiti di intervento prioritari sono stati non soltanto le riforme dei processi e dei riti che abbiamo di recente varato in quest'Aula, ma anche gli interventi di modifica al codice dell'insolvenza, che ci ha occupato particolarmente in questo approfondimento. È fondamentale pertanto, con specifico riguardo all'ultimo degli obiettivi richiamati, in particolare negli allegati al PNRR, apportare le modifiche evidenziate al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, attuando quindi in maniera molto chiara e del Consiglio europeo, relativa alle procedure di ristrutturazione, esdebitazione e insolvenza. Si devono quindi rivedere gli accordi di risoluzione extragiudiziale, al fine di incentivare le parti a farne un maggior uso, anche in un'ottica deflattiva e di snellimento, potenziando i meccanismi di allerta; specializzando gli uffici giudiziari e le autorità amministrative competenti per le procedure concorsuali; implementando la digitalizzazione delle procedure, anche attraverso la creazione di un'apposita piattaforma *online*, tema assolutamente da sviluppare. Chiaramente questo è l'esito

nonché a eliminare ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali, su cui tanto ci stiamo battendo, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e le procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva,

Signor Presidente, gli effetti della pandemia ancora si riscontrano e si riscontreranno per molto tempo nell'ambito della situazione economica del nostro Paese, in particolare sulla funzionalità delle imprese. Pertanto, condivido l'iniziativa del Governo di aver rinviato l'entrata in vigore del decreto legislativo del 2019 e di aver introdotto degli strumenti che possono aiutare a risolvere i problemi delle imprese e che non potevano essere affrontati con gli istituti della legge fallimentare. Devo dire, signor Sottosegretario, che condivido tutto della nuova legge, come dirò tra poco.

della soluzione di problemi urgenti della giustizia. Tutti sappiamo che l'esame per avvocato si svolge i primi di dicembre e, quindi, non aver tenuto conto che quella normativa poteva essere inserita in questo decreto-legge - a mio avviso - è stato un errore.

«opera in modo professionale, riservato, imparziale», il che vuol dire che non avrà la necessità di ricorrere a pubblicità, conferenze stampa e cose del genere, ma l'intento è dare imparzialità alla sua funzione.

Credo che fosse necessario introdurre un elemento che variasse a seconda del soggetto che doveva essere nominato, prendendo spunto dalla sede dell'impresa, al fine di indicare un quarto membro che fosse indicato dal presidente del tribunale o dal presidente della sezione fallimentare, per avere contezza della situazione politica, economica e sociale di quella determinata zona.

alla questione dell'esperto, dovrò perdere qualche minuto, perché mi rendo conto ogni giorno di più

Per fare un esempio, anche prendendo spunto dalla mia posizione, io svolgo la funzione di senatore, ma contemporaneamente anche quella di presidente della commissione contenziosa.

Come senatore, svolgo la mia attività tenendo conto della politica, delle mie idee, delle politiche del mio partito, del mio Gruppo parlamentare e sviluppo un'azione politica in quel senso. Le due questioni sono in contrapposizione? No. Quando mi trovo a giudicare dei vitalizi, da giudice devo dire se la legge è stata o meno violata;

Il giudice, però, deve garantire la certezza del diritto, come l'esperto che andiamo a nominare deve avere quella professionalità forte che gli consente di resistere a qualsiasi indicazione gli venga da coloro che l'hanno nominato.

ma ricorrevano all'amministrazione controllata per risolvere e salvaguardare la residua capacità occupazionale dell'azienda.

nella gestione delle attività imprenditoriali. In effetti su questa parte i relatori hanno modificato in meglio la lettera iniziale del provvedimento, che addirittura distingueva tra professionalità e so che anche il Sottosegretario è stato

un esperto che deve portare per forza alla salvezza dell'azienda? No. Se è un vero esperto e professionalmente preparato, nel momento in cui si accorge dell'impossibilità di arrivare alla salvezza dell'azienda, deve rinunciare e far sì che possa essere archiviata la domanda. Questa è la logica

e noi l'abbiamo scritta per rendere un servizio al Paese. In un momento di difficoltà vogliamo dare un effettivo ausilio all'impresa ma, nello stesso tempo, anche un contributo che sia tale da non disperdere soldi inutili al fine di realizzare il massimo dell'occupazione possibile e superare le difficoltà del momento. *(Applausi)*.

Il primo è stato quello del rinvio dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ad eccezione delle parti relative alle procedure di allerta e alla composizione assistita della crisi innanzi all'organismo di composizione della crisi d'impresa (Ocri),

cui si accede tramite una istituenda piattaforma telematica nazionale, che offre all'imprenditore l'affiancamento di un esperto terzo e indipendente per agevolare, in maniera anche riservata, le trattative con i creditori.

possiamo provare a sviluppare un ragionamento anche dal punto di vista della crisi di impresa. Il provvedimento apporta tutta una serie di modifiche alla legge fallimentare - ecco perché attiene di più all'ambito della giustizia - con l'anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale previsti dal codice della crisi. Il lavoro che abbiamo svolto in sede di Commissione ha cercato di migliorare, per quello che è stato possibile, il provvedimento. Per questo ringrazio il sottosegretario Sisto

È stato un lavoro proficuo e di sinergia, che insieme abbiamo svolto, in particolare con l'approvazione di alcune proposte che prevedono che la piattaforma venga gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico. un intervento sulle modalità di iscrizione nell'elenco degli esperti; l'inserimento di specifiche disposizioni in materia di procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi; la proroga della data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022 e del termine temporale per la prima nomina del revisore o degli organi di controllo da parte di talune società a responsabilità limitata e società cooperative; la garanzia che l'esperto sia un soggetto non legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento dei rapporti di natura personale e professionale; e molte altre modifiche modifiche che andranno ulteriormente migliorate nel testo del provvedimento. Segnalo, in particolare, l'accoglimento dell'ordine del giorno già presentato dal mio Gruppo volto ad estendere, di seguito agli esiti del monitoraggio da eseguire dopo dodici mesi dalla data di operatività della piattaforma, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con sede nel distretto di ciascuna corte d'appello con tribunale sezione imprese, la formazione dell'elenco degli esperti, il luogo in cui la domanda di iscrizione nell'elenco deve essere presentata e il sito in cui la commissione che nomina l'esperto deve avvenire. Con questo ordine del giorno si vuole porre rimedio a una anomalia che potrebbe di fatto mettere in difficoltà le imprese di alcune aree del Paese che, avendo un'alta densità di imprese iscritte, rischierebbero fortissime difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi che il provvedimento si prefigge. Ci abbiamo provato da questo

impegna il Governo a valutare la possibilità di specificare, con apposito provvedimento normativo, le modalità e i requisiti di partecipazione delle associazioni di categoria del livello locale. Mi piace, inoltre, porre l'attenzione anche sull'approvazione di un nostro emendamento, che prevede che le disposizioni in esame si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il turismo generato da questo comparto è quello sostenibile socialmente, legato in particolare alla rete International youth hostel federation, che, avvalendosi dell'esperienza dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, fondata nel dicembre 1945, consente a molti di godere dei 1.154 siti UNESCO sparsi nel nostro Paese. avvio a concludere. Quanto descritto si colloca nel percorso di rinascita del nostro Paese e di rafforzamento del tessuto delle nostre imprese, che questo Governo cerca di proporre. Abbiamo assistito nell'appena trascorsa stagione estiva un notevole incremento del lavoro e del fatturato; vengo da una provincia turistica e, quindi, ho vissuto con mano tale incremento. Questo

considera veramente la riforma della giustizia come una infrastruttura orizzontale che interessa tutti i settori di intervento dello stesso Piano. Anch'io mi approccio in maniera favorevole favorevole all'analisi del provvedimento che ci apprestiamo a votare e soprattutto a una serie di istituti che vanno veramente nella direzione della velocizzazione e della semplificazione. - ad esempio - alla composizione negoziata della crisi, l'istituto volontario al quale possono aderire gli imprenditori sapendo di essere affiancati da professionisti. Ha ragione il collega Caliendo quando afferma che

sappia svolgere un'analisi effettivamente concreta, positiva, volta non solo a ristrutturare il debito - certamente è un tema sul quale va posta una grande attenzione - ma anche soprattutto a riposizionare l'azienda su nuovi mercati, verso nuovi clienti, su nuove politiche commerciali e così via. Non è detto, cioè, che questi professionisti sappiano bene come riallocare i fattori produttivi all'interno dell'azienda. Quindi, si spera proprio che abbiano nel loro *skill* queste competenze, perché le altre sono le cosiddette competenze di base, quelle sulla base delle quali i commercialisti e gli avvocati già assistono noi imprenditori. Riconvertire un'azienda su un nuovo paradigma commerciale, su nuovi mercati, è, invece, azione molto più complessa che richiede la capacità tipicamente imprenditoriale - su questo potremmo aprire una

nonché di saper allocare bene - ripeto - questi fattori produttivi, che sono sia le risorse umane con le loro qualificazioni, le loro professionalità e i loro ruoli sia i capitali finanziari.

e, quindi, portare un'analisi di carattere economico-aziendale più che un'analisi che interpreta - anche perché, sono molto sincera e devo dire che non sono in grado di farlo - gli strumenti giuridici a disposizione. Un sistema efficiente di gestione delle crisi di impresa è - come sappiamo tutti - un fattore davvero molto importante per lo sviluppo di un Paese, perché l'evoluzione delle conoscenze e del contesto socio-economico modifica moltissimo il quadro competitivo, al punto che potrebbe ribaltare anche un ordine di priorità all'interno dei settori.

questi cambiamenti, davvero molto veloci e repentini, tipici dell'epoca che stiamo vivendo, impongono anche la capacità di intercettare

dalle aziende che invece potrebbero avere un debito meno importante e molto più semplice da ristrutturare, ma che non hanno al loro interno quei fattori produttivi in grado di intercettare le nuove sfide. Se si sbaglia questa distinzione, in un contesto in in un contesto in cui ci sono strumenti che agevolano l'interlocuzione dell'imprenditore con il suo professionista di fiducia per gestire un momento di crisi e riportare l'azienda nella competizione economica, si rischia di salvare tutte le aziende. Quindi la mia raccomandazione è certamente di avere

i fattori produttivi, ma soprattutto le risorse umane e, di conseguenza, il vero problema del nostro Paese, che è il ricambio generazionale. Abbiamo una serie di piccole e medie imprese a conduzione familiare in cui, come sapete, il ricambio generazionale rappresenta

pari ad 1,5 miliardi di euro, non solo per introdurre la formazione digitale, ma anche per la formazione finanziaria nelle scuole. Ciò è molto importante, perché credo che in Italia ci siano due analfabetismi: quello digitale e quello finanziario. La leva finanziaria

dedicarsi a rilanciare le imprese e comprendere il *business* di ogni singolo imprenditore, devono impiegare le loro risorse - che, lo ripeto, sono estremamente costose - in queste procedure per risolvere le crisi.

quindi nel merito dei problemi perché non sono uso scapparne, ma certamente sono anche solito ricordare le affermazioni poco democratiche che vengono pronunciate in questi giorni, in un clima nel quale il confronto civile dovrebbe essere dimostrato prima di tutto da chi ha incarichi politici e ricopre ruoli importanti e di riferimento per il nostro Paese.

Qualche aiuto si doveva e si poteva dare ai settori più colpiti dalla crisi e dalla pandemia. Si poteva affrontare anche il tema del credito, perché sappiamo - o, meglio, dovrebbe sapere chi è uso a impegnarsi professionalmente nelle aziende italiane - che il credito è uno dei temi fondanti e fondamentali della crisi d'impresa.

credito. Tra pochi giorni, alla fine di questo mese, avremo la completa attuazione di Basilea 3, con ulteriori difficoltà per dare liquidità e credito alle nostre imprese.

Abbiamo cercato di avanzare delle proposte, come è consuetudine di un partito assolutamente all'interno dell'arco costituzionale, di un partito, cari colleghi del Partito Democratico, che sta difendendo da solo, con un piccolo manipolo di valorosi

Mi piacerebbe rileggere agli amici del MoVimento 5 Stelle quello che dicevano nella scorsa legislatura sul ricorso al voto di fiducia; mai come in questa legislatura, nella quale siete stati al Governo con tutte le maggioranze possibili,

abbracciate e ieri offendevate. Mi piacerebbe capire chi è che sta lottando contro l'abuso della decretazione d'urgenza, chi è che sta cercando di difendere la libertà dei cittadini di non dover sottostare a un *green pass* obbligatorio (unico Paese al mondo),

Colleghi, Fratelli d'Italia non finirà di difendere le libertà e di difendere la Costituzione, che quelli che si ritengono all'interno dell'arco costituzionale stanno tradendo ogni giorno. Non si fermerà di fronte a nulla e continuerà a difendere gli italiani, a difendere i cittadini e i lavoratori. Abbiamo anche presentato un emendamento importante, che non aveva colore politico, non era né di destra, né di sinistra. è stato semplicemente dichiarato inammissibile. Credo che sia giusto che si sappia che Fratelli d'Italia chiedeva, se aveste accolto il nostro in cassa integrazione senza possibilità di continuità dell'attività, perché magari in cassa integrazione a zero ore di imprese fallite, potessero

Ebbene, sì, ce lo avete reso inammissibile; voi avete reso inammissibile un provvedimento che noi chiedevamo per facilitare l'assorbimento nell'economia reale di quei lavoratori - ribadisco - in cassa integrazione a zero ore e senza possibilità di avere avere un futuro. La maggioranza, il Governo, la Presidenza del Senato lo ha dichiarato inammissibile. E questo nasce non da intuizioni, ma nasce dalla conoscenza dei problemi delle aziende, nasce dal fatto che nel mio Trentino un'azienda che dà lavoro a 100 dipendenti rischia di chiudere perché l'INPS le sta contestando i benefici del Jobs Act, dopo che loro avevano salvato lavoratori a zero ore in cassa integrazione. Allora, colleghi, sui temi confrontatevi e non chiudetevi all'interno delle barriere e degli steccati. Evitate di fare quello che sta succedendo ignobilmente in queste ore, dove, invece che parlare delle imprese, delle aziende e dei problemi di Torino, di Milano e di Roma,

tentativo di andare incontro alle tante imprese che nel nostro Paese si trovano in situazione di crisi incolpevole. Tutti noi che lavoriamo sul territorio e che conosciamo le imprese del nostro splendido Paese sappiamo quanto la crisi originata dal Covid, ma prima ancora la crisi economica, avesse provocato nel tessuto imprenditoriale profonde lacerazioni e molto spesso

Tutte le soluzioni per una composizione negoziata della crisi di impresa ci vedono favorevoli, come favorevoli ci vedono tutte le figure professionali che vanno ad affiancare l'imprenditore nel momento della sua difficoltà. A tal proposito, vorrei soffermarmi brevemente sulla peculiarità del tessuto imprenditoriale italiano che molto spesso è composto da piccole e medie imprese di stampo familiare. Si tratta di aziende che non licenziano, che non vanno in cassa integrazione, ma che semplicemente aggiungono un buco alla cintura

ma sono sicuro che il sottosegretario Sisto era attento perché con noi ha lavorato in modo alacre per migliorare il testo,

chiede cassa integrazione perché il dipendente è normalmente il figlio, il nipote, la nuora, la moglie e il marito. marito. Questo tessuto, che da legame e sodalizio di vita diventa anche legame e sodalizio economico, capace di arricchire di far crescere la nostra economia, è prezioso e noi in questa Aula abbiamo il compito di proteggerlo e difenderlo. La piccola, media e anche grande impresa familiare ha dato lustro al nostro Paese e ha trasformato, come ben sappiamo, i distretti i distretti produttivi in un modello che viene studiato in tutto il mondo. La norma cerca allora di offrire all'imprenditore che si trova in crisi incolpevole un aiuto e un soccorso che non siano quelli del fallimento o il classico portare i libri in tribunale, come purtroppo fino ad oggi sostanzialmente è stato, ma si identifica e si va a inventare la figura dell'esperto si pone in una situazione in cui può non solo consigliare, ma anche proteggere

una norma, quanto mai provvida, che rimette al centro anche il compito delle camere di commercio che sono, a loro volta, una eccellenza del nostro Paese e che con questa norma vengono valorizzate. L'unico L'unico piccolo appunto è la speranza che il nostro ordine del giorno, che è stato accolto dal Governo, diventi poi realtà e si permetta non solo alle camere di commercio dei capoluoghi di Regione, ma anche alle camere di commercio delle città sede di corte di appello di poter intervenire in modo efficace a sostegno delle aziende del loro territorio, attraverso un coinvolgimento diretto nei meccanismi previsti dalla norma. Dico questo perché ho presente l'esempio della mia città natale, Brescia, che è capoluogo di Provincia, sede di corte d'appello, al centro di un distretto industriale tra i più floridi del nostro Paese e che però, *rebus sic stantibus*, dovrebbe fare riferimento a Milano per tutto quanto riguarda le procedure previste da questa norma. La stessa cosa accade però a Lecce, altro centro di

mira a monitorare la situazione con l'impegno di rivederla tra un anno, come il sottosegretario Sisto ci ha garantito, per verificare l'opportunità di estendere anche ai capoluoghi di Provincia, sede di corte di appello, tutto quanto previsto oggi solo per le camere di commercio dei capoluoghi di Regione. In conclusione, Presidente, cari colleghi, dobbiamo continuare su questa strada. La strada non può essere quella di avere, da una parte, un aumento della fiscalità, cosa assolutamente esecrabile e non accettabile e, dall'altra, una sorta di abbandono a se stesso del tessuto imprenditoriale. Dobbiamo risollevare, sostenere e valorizzare le sorti di chi oggi - uso una parola forse eccessiva, ma spero non lo sembri - eroicamente ancora si mette a fare impresa, eroicamente ancora decide di dare lavoro,

ma che deve essere completato dal più grande e più importante dei tasselli che è quello, da una parte, della semplificazione burocratica e, dall'altra, della semplificazione e dell'alleggerimento fiscale. Queste due misure sono indispensabili, perché non vorrei dimenticassimo in questa sede che, molto spesso, gli imprenditori vanno in crisi perché è lo Stato che non paga. Non accada mai più che un imprenditore si trova in crisi perché lo Stato non paga. È qualcosa che noi, in quest'Aula, non possiamo permettere. Ringrazio i colleghi che, sia in Commissione sia in Aula, hanno votato e voteranno per questo decreto che, come ho detto, è un passo nella giusta direzione, ma è un piccolo passo. Per sostenere le nostre imprese sul piano internazionale, sul piano della ormai totale globalizzazione economica e imprenditoriale, dobbiamo fare ancora molto, ma molto di più.

è stata da sempre al centro dell'azione politica del MoVimento 5 Stelle. Si tratta di un principio generale che ha animato la nostra attività dentro e fuori le aule parlamentari. Un principio che valeva già prima che la pandemia travolgesse il mondo intero e il nostro Paese e che vale ancora di più adesso, che stiamo finalmente uscendo dal periodo più buio della pandemia. Questo rappresenta per noi un concetto *omnibus*, che certamente va applicato a cittadini e lavoratori, ma anche e soprattutto alle nostre imprese. In questi mesi un dato è apparso molto chiaro: se si ferma il nostro tessuto produttivo, si ferma il Paese. Diverse volte sono intervenuto in quest'Aula per sottolineare l'importanza di superare velocemente e con decisione la fase più acuta della pandemia, permettendo alle nostre imprese di tornare a correre e a trainare l'economia. Soprattutto con il precedente Governo Conte, siamo riusciti a mettere in piedi un sistema che garantisse a imprese, lavoratori e professionisti ristori in tempi brevi; ma eravamo e siamo consapevoli che il miglior sussidio che lo Stato può dare all'intero tessuto produttivo è soprattutto quello di garantire le migliori condizioni possibili per favorire la crescita e la continuità delle imprese e per favorire la nascita di nuove. Nella primavera 2020, durante la fase più acuta della pandemia, non abbiamo mai abbandonato il nostro tessuto produttivo. Col decreto cosiddetto Cura Italia prima e col decreto liquidità poi, abbiamo messo a regime un imponente meccanismo per dare alle nostre imprese il sostegno necessario, meccanismo che poi è stato oliato e rimesso a punto per tutti i mesi della pandemia. Con il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e soprattutto con il piano Transizione 4.0, abbiamo innalzato il livello. Lo ripetiamo da tempo: aiutare le aziende che decidono di investire, *in primis* su se stesse, deve essere sempre una priorità e per noi del MoVimento 5 Stelle questo principio ha sempre rappresentato una stella polare della nostra azione politica, con buona pace di chi per anni ci ha bollato, in maniera sconsiderata, come forza politica anti imprese. Non solo: per i crediti di imposta di Transizione 4.0, siamo convinti che si debba ragionare al più presto sull'opportunità di renderli cedibili, in maniera tale da dare una ulteriori iniezione di liquidità alle nostre aziende e favorire investimenti consistenti. Insomma, un superbonus imprese, sulla scia dei grandissimi effetti benefici che sta avendo per il comparto dell'edilizia il superbonus al 110 per cento. Su questa misura, in tanti in origine avevano sollevato perplessità e dubbi, ma i numeri ci dicono che l'insistenza del MoVimento 5 Stelle aveva e ha la sua ragione d'essere. Giusto ieri, il Consiglio nazionale degli ingegneri, studiando i *trend* dei primi nove mesi dell'anno, ha stimato, per fine anno, impegni di spesa per 9,5 miliardi, con un valore aggiunto di oltre 19 miliardi ed effetti sul PIL per 12 miliardi. La stima più interessante riguarda, però, i nuovi posti di lavoro: 153.000, tra indiretti e diretti. Se pensiamo alle condizioni in cui versava l'intera filiera solo due anni orsono, verrebbe da dire che il superbonus ha consentito a un intero segmento della nostra economia di risorgere. Per questo insistiamo tanto sul prolungamento dell'incentivo, magari con un orizzonte pluriennale e non solo fino a tutto il 2023, come del resto hanno chiesto ieri gli ingegneri italiani. Lo Stato deve dunque seguire e accompagnare l'intera vita delle aziende, sostenendole nei momenti di maggiore prosperità, con l'obiettivo di agevolarne gli investimenti e l'espansione, ma anche e soprattutto nei momenti di fisiologica flessione economica. Il provvedimento prende le mosse da quest'ultima necessità, introducendo in favore delle imprese gli strumenti incentivanti per la ristrutturazione o il risanamento aziendale. In primo luogo viene differita ulteriormente l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa fino a maggio 2022. La corposa novella era stata pensata per rinnovare l'ordinamento nel 2019, in un contesto che non poteva tenere conto dei devastanti effetti della pandemia. Pertanto si rende necessaria una doverosa riflessione su tale intervento riformatore, alla luce delle nuove esigenze sorte negli ultimi mesi e soprattutto per gli effetti che rimarranno anche a pandemia conclusa. *Medio tempore*, tuttavia, abbiamo deciso di recepire sin d'ora nell'attuale tessuto normativo previsto dalla cosiddetta legge fallimentare, alcune disposizioni contenute all'interno del codice della crisi d'impresa, come la disciplina relativa agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, *ex* articolo 182-*septies,* che troverà applicazione a tutte le categorie di creditori, eliminando la limitazione precedentemente in essere ai soli creditori e intermediari finanziari. Il decreto-legge prevede anche la modifica della disciplina della convenzione in moratoria (nuovo articolo 182-*opties*), estesa a tutte le categorie di creditori. Viene inoltre previsto l'istituto degli accordi di ristrutturazione agevolati (articolo 182-*novies*), che permette di concludere un accordo di ristrutturazione dei debiti con una soglia di creditori aderenti dimezzata, del 30 Il decreto-legge mira anche a sostenere le imprese in crisi e a favorire il risanamento aziendale. In questa direzione è stato introdotto il nuovo istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa. In breve, a partire dal 15 novembre prossimo gli imprenditori che si troveranno in condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario e che quindi rischiano una crisi o di rendersi insolventi, al fine di avviare proficuamente il risanamento aziendale potranno richiedere al segretario generale della camera di commercio di riferimento la nomina di un esperto indipendente. Tale soggetto avrà il compito di agevolare le trattative tra tutti i soggetti coinvolti (imprenditore, creditori ed eventuali altri soggetti interessati), con l'obiettivo di individuare una soluzione per superare lo stato di crisi. A conclusione della procedura di composizione negoziata sono previste altresì anche importanti misure premiali per l'impresa, come la riduzione degli interessi sui debiti tributari, la riduzione al minimo delle sanzioni e la possibilità di ottenere un piano di rateizzazione delle somme dovute. Infine, ma non in ordine di importanza, ho il piacere di segnalare anche la norma introdotta nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite 2a e 10a, che autorizza un nuovo bando per l'assunzione di 500 magistrati ordinari, da svolgersi secondo modalità in grado di garantire la celere conclusione della procedura selettiva, prestando massima attenzione alla valutazione dei candidati più meritevoli. Ritengo sempre positivo quando in quest'Aula si dibatte su temi di stretto interesse per le nostre imprese, anche nel caso in cui si tratti di interventi di elevata e particolare complessità tecnica. Gli incoraggianti dati sulla ripresa economica devono spingerci a fare ancora di più. Come ho già detto prima, l'impatto che il superbonus al 110 per cento è riuscito a dare all'intero indotto dell'edilizia deve costituire un esempio virtuoso cui fare costante riferimento, al fine di convincere l'intero emiciclo parlamentare dell'importanza ormai indifferibile di puntare su misure altamente incentivanti anche in altri settori, che siano in grado di favorire la crescita economica delle imprese e quindi dell'intero Paese, perché, come ho detto poc'anzi, se ripartono le imprese, riparte l'Italia.

ho ascoltato con attenzione i colleghi, che hanno confermato il lavoro che è stato fatto, insieme al sottosegretario Sisto, che vedo, e al sottosegretario Bini. Li vogliamo ringraziare per il

che naturalmente sono anche il frutto della scelta che ha fatto il Parlamento per cercare di offrire delle spalle molto larghe al Paese, considerando il periodo che stiamo attraversando.

lo hanno detto i colleghi e lo ha detto anche il relatore Collina con molta chiarezza nella sua relazione, ci aspetta

abbiamo portato avanti il provvedimento, alla sottosegretaria Bini e al sottosegretario Sisto e ai colleghi delle Commissioni riunite. Voglio solo aggiungere una considerazione: durante le audizioni che abbiamo svolto per la conversione di questo decreto-legge abbiamo potuto registrare la consapevolezza di tutte le associazioni di categoria,

È un fatto importante, perché credo che sia le categorie professionali che le associazioni di impresa avranno un ruolo importante nel dare

che una volta tanto non è di stile, ma dà atto dell'impegno dei relatori e di tutti i parlamentari in Commissione - ma per ribadire che questo provvedimento si colloca nell'ambito di un *new deal* delle scelte dei rapporti fra Stato e imprese, fra procedure ed esperienze, perché in realtà stiamo coniando progressivamente, con uno sforzo sinergico, non più un diritto dell'impresa, ma un diritto per l'impresa. Il tentativo è quello di ragionare in modo diverso, perché l'impresa oggi non è più un oggetto di verifica *tout court*, un punto di riferimento importante per la ripartenza: in questa logica, il provvedimento in esame si colloca in perfetta assonometria sia con la riforma del processo penale, sia con la riforma del processo civile, in cui gli istituti premiali devono fare certamente i conti con un passato che non è che venga ripudiato, ma viene riletto in una considerazione realistica del momento che stiamo vivendo. Mi sembra quindi che questo provvedimento sia un altro tassello importante, che costituisce per questo Governo il riconoscimento effettivo di come si possa far ripartire un Paese con una sola parola: riconciliazione.

Signora Presidente, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-*ter*, del Regolamento del Senato, il testo di un emendamento che recepisce integralmente le proposte emendative approvate dalle Commissioni riunite, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, sul quale, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, intende porre la questione di fiducia.

pertanto lo trasmette alla 5a Commissione. Ai sensi dell'articolo 102-*bis*, la Commissione bilancio è autorizzata a convocarsi. Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2371,

Come già stabilito e concordato dalla Conferenza dei Capigruppo, le dichiarazioni di voto avranno luogo domani mattina. *(Reiterati

quale permangono delle opacità. Attilio Manca era un giovane urologo di Barcellona Pozzo di Gotto, con davanti una brillante carriera, legato pertanto alla prostata di un *boss* mafioso, Bernardo Provenzano, e perciò assassinato nel lontano 2004. Che colpa ha avuto il nostro Attilio, se non quella di essere originario di Barcellona in Sicilia e di avere come cugino Ugo Manca, molto amico di Angelo Porcino, esponente mafioso di Barcellona, un luogo di capitale importanza nella geopolitica mafiosa degli anni Ottanta fino ai primi anni del 2000? ringraziare la protervia dei familiari, della madre, Angela Gentile, e dell'avvocato Fabio Repici, che ha così bellamente portato avanti la ricerca della verità sul delitto di Attilio. È un delitto che ha tutte le caratteristiche di quello mafioso,

laddove i suoi amici di infanzia, siciliani, riferirono che aveva una certa frequenza con la droga. Lo ricordo, dunque: Barcellona Pozzo di Gotto, un paese ad alta densità mafiosa, contro l'idea dei suoi colleghi medici di Viterbo, con cui lavorava fianco a fianco. Ci sono troppe opacità nel suicidio-omicidio di Attilio Manca: una volta chiarite, ci darebbero un'immagine più realistica della nostra società e dello stato di salute della nostra democrazia. L'assassinio di Attilio ci darebbe elementi di conoscenza sulla trattativa Stato-mafia, che da sempre, almeno dalla nascita della nostra Repubblica, hanno connotato la nostra storia nazionale e l'anomala storia di quanto accaduto, a partire dalla strage di Portella della Ginestra, fino a quelle di via Fani, con il delitto Moro, di Capaci e di via D'Amelio.

raccapricciante sentirle dire che è stata pure privata della cura del giardino di casa, perché le hanno avvelenato le piante. Questo è quanto emerso dall'analisi sul terreno: piante avvelenate da un diserbante fuori commercio (Roundup). Perché poi l'allora presidente della Repubblica Napolitano chiamò la procura di Viterbo - fatto emerso durante la conferenza stampa a Viterbo di Petroselli e Pazienti,

Nessuno dei 31 progetti finalizzati al miglioramento della gestione delle risorse idriche a uso irriguo (per 422 milioni di euro) è risultato ammissibile per motivi tecnici. I progetti presentati dalla Regione, infatti, non rispettavano alcuni dei 23 criteri stabiliti dall'Unione europea, che dovevano invece essere tutti soddisfatti. Addirittura uno dei progetti presentati era già stato finanziato in precedenza, mentre 17 prevedono una durata di intervento e realizzazione delle opere oltre i trenta mesi, limite massimo dettato dallo stesso PNRR. Parliamo di criteri che le Regioni italiane conoscevano bene, visto che mesi fa il Governo aveva condiviso con le stesse i parametri di ammissibilità e aveva anche attivato un servizio di assistenza tecnica per fornire chiarimenti ed evitare errori materiali. La responsabilità di questa bocciatura è quindi della Regione Siciliana e, come molti siciliani, anch'io sono rimasto sconcertato per tale ingiustificabile errore. Per anni, infatti, ci siamo sentiti dire che mancavano le risorse economiche necessarie a realizzare i progetti di ammodernamento delle reti idriche. Adesso, invece, abbiamo la dimostrazione che la Regione è priva di programmi di intervento e di azione efficaci a risolvere in tempi brevi l'annoso problema dell'acqua. Ora bisogna trovare urgentemente una soluzione affinché la Sicilia non perda questi finanziamenti, con il contributo di tutti e senza polemiche, selezionando i progetti che si prestano a correzioni, modifiche o rimodulazioni, concordando gli interventi con gli organi tecnici del Ministero e condividendo il risultato con il ministro Patuanelli, che proprio domani incontrerà l'assessore regionale all'agricoltura Scilla. A tal proposito, intervenuto alla Camera, il Ministro ha precisato che la Sicilia non sarà lasciata sola. Nel PNRR, infatti, ci sono 880 milioni a sostegno del sistema agricolo per l'acqua a uso irriguo, mentre altri 440 milioni sono previsti dalla legge di bilancio e non soggetti alla tempistica del Piano. Pochi giorni fa il professore Andrea Guerrini, componente del collegio di ARERA, ha ben fotografato il momento. La sfida più urgente è al Sud: serve un'azione decisa del legislatore per risolvere inadempienze nella creazione degli enti d'ambito che influiscono sul servizio idrico e sulle agevolazioni agli utenti. Colleghi, dobbiamo essere pronti per affrontare le sfide che questo tempo ci impone e non possiamo permetterci fallimenti come quello compiuto dalla Regione Siciliana. Questo è il momento della politica e delle decisioni giuste. La Sicilia non può perdere altre importanti occasioni di sviluppo: sarebbe imperdonabile.

gli ambiti territoriali provinciali e gli uffici scolastici regionali sarebbero incorsi in numerosi errori. La procedura informatizzata utilizzata per l'attribuzione e la valutazione dei punteggi del personale precario avrebbe generato una serie di inesattezze, con conseguenti penalizzazioni. Roma risulterebbe la città più colpita da questo abuso. Tale problematica avrebbe determinato ad oggi, solo nel Lazio, l'assenza di circa 3.600 docenti di ogni ordine e grado. In alcune Regioni, l'algoritmo è rientrato recuperando alcuni candidati esclusi dalla prima tornata, seguitando lo scorrimento della graduatoria in modo casuale e in altri casi no. Il sistema informatico messo a punto dal Ministero non avrebbe quindi seguito un procedimento valido e corretto, non considerando il punteggio posseduto da ogni aspirante docente in graduatoria. Sarebbero pochissimi i docenti in Gae individuati sia nel primo sia nel secondo bollettino nomine; sarebbero stati individuati in entrambi i bollettini docenti con punteggio e posizioni bassissime, a discapito pertanto di altri con punteggio e posizioni più favorevoli. Sarebbero stati individuati docenti su classi di concorso a loro non spettanti; moltissimi sarebbero considerati rinunciatari, nonostante le scuole scelte in fase di domanda e nonostante avessero comunicato i posti dell'ambito territoriale provinciale, il quale ora imputerebbe addirittura a loro stessi Moltissimi insegnanti che avrebbero prodotto reclamo avverso il primo bollettino, ad oggi non avrebbero ottenuto risposta, risultando ancora una volta esclusi. L'algoritmo avrebbe ripreso a convocare l'ultimo nominato del primo bollettino e avrebbe portato in cattedra niente meno che gli studenti dell'ultimo anno. Si evidenzierebbero il mancato riconoscimento dei titoli di riserva e mancate nomine su cattedre di sostegno. Si riscontrerebbe anche il conferimento di cattedre in sede non indicata in domanda, non rispettando la graduatoria delle sedi indicate, a vantaggio di un altro aspirante peggio graduato. starebbe mettendo in pericolo l'ordinario svolgimento delle attività curriculari, con inevitabili ricadute sull'apprendimento degli studenti. Nell'attuale e persistente situazione pandemica emergenziale, le istituzioni scolastiche sono fra le categorie più coinvolte per un sereno ritorno alla normalità in favore di tutti gli studenti. Prendere in esame ciò che si starebbe verificando potrebbe garantire di fatto alle scuole un'organizzazione più adeguata e un migliore funzionamento.

DISEGNO DI LEGGE Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia